L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che, come da accordi intercorsi tra i Gruppi, la discussione delle mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR, già in calendario per giovedì 22 giugno, sarà anticipata al pomeriggio di domani, dopo la commemorazione del senatore Berlusconi. I tempi della discussione prevedono cinque minuti per l'illustrazione e quindici minuti a ciascun Gruppo, ripartibili tra discussione e dichiarazione di voto. La terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, già prevista per martedì 27 giugno, è rinviata ad altra data,

non si è potuto svolgere in maniera compiuta a causa del sopraggiungere del termine in scadenza costituzionalmente previsto per la decretazione d'urgenza.

certamente i tempi della prima lettura parlamentare, ma affrontando un lavoro eccezionale, molto accurato e impegnativo, svolto in maniera corale e collaborativa dai colleghi delle Commissioni lavoro e affari costituzionali della Camera. colleghi - deve necessariamente essere convertito in legge entro il 21 giugno e per tale ragione, rilevato anche l'elevato numero di emendamenti presentati (241 emendamenti e 70 ordini del giorno), le Commissioni riunite 1a

in relazione a quanto riferito dal senatore Zaffini, il disegno di legge n. 747, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44,

si tratta di un provvedimento che si occupa molto poco dei problemi strutturali della pubblica amministrazione, a partire dalla carenza dell'organico, dalla precarietà - ci sono tanti precari nella nostra pubblica amministrazione - e dai rinnovi contrattuali. Non c'è traccia di questi problemi, che richiederebbero invece risposte concrete e immediate. Non c'è traccia di quel rafforzamento che viene richiamato nel nome che porta con sé questo sé questo decreto-legge. Ci si limita a interventi *spot* senza futuro e senza una strategia per il comparto. Prima di entrare nel merito del provvedimento, non si può non evidenziare negativamente l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza parlamentare nell'*iter* di conversione in legge del decreto. Alla Camera il Gruppo Partito Democratico ha cercato di correggere molte storture del testo e di andare incontro alle risposte richieste dal comparto. Ma, tranne alcune rare eccezioni, è stata registrata una chiusura totale; ancor peggio al Senato, dove questo decreto è arrivato in tutta fretta, senza possibilità di confronto in Commissione, con tempi ristrettissimi per la presentazione degli emendamenti. Il risultato è che il disegno di legge è arrivato in Aula senza relatore, a dimostrare un atteggiamento di scarso interesse a un confronto produttivo. Vengo al merito del provvedimento in esame. La pubblica amministrazione è sotto organico, con molti contratti a termine e stipendi che non sono minimamente allineati all'inflazione: una situazione che richiederebbe interventi strutturali e un'attenta programmazione pluriennale. Con questo disegno di legge, invece, siamo davanti a un piano di assunzioni del tutto inadeguato, anche solo per colmare i prossimi pensionamenti, figuriamoci poi per far fronte alle grandi sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da qui al 2026. Insomma, niente è stato fatto a proposito dei precari storici della pubblica amministrazione, che sono in gran parte nel settore sanitario; niente sul rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024, esattamente come nulla era previsto nel DEF. Niente è stato fatto per un piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, che avrebbe dovuto sostenere l'attuazione del PNRR. I nostri emendamenti andavano esattamente in quella direzione, è sbagliato l'approccio generale. Non si può riformare la pubblica amministrazione pensando solo agli assetti di vertice, senza intervenire su chi ogni giorno, nei vari settori, porta avanti il proprio lavoro. Nonostante nel 2026 siano previsti comunque 300.000 dipendenti in meno, che saliranno a 700.000 nel 2030; nonostante il vuoto normativo lasciato dalla recente legge di bilancio sul rinnovo dei contratti collettivi; nonostante il 15 per cento dei lavoratori nella pubblica amministrazione sia attualmente precario, il Governo ha precluso ogni iniziativa nel merito riguardante un aumento dei diritti dei lavoratori e nuove assunzioni. Le assunzioni di cui si parla nel provvedimento riguardano prevalentemente le Forze di polizia: assunzioni utili e necessarie, ma insufficienti nei numeri e nei comparti interessati dall'uscita dei dipendenti per raggiunti limiti di età. L'Italia registra ad oggi il dato più basso nel rapporto tra numero di residenti e lavoratori pubblici, con una percentuale del 5,6

Serve una stabilizzazione di queste figure che svolgono già da anni nella pubblica amministrazione funzioni delicatissime. Il riferimento è agli uffici per il processo, alle prefetture, alle agenzie per la coesione, dove i lavoratori precari assicurano il buon funzionamento dello Stato.

per lavorare in uffici molto delicati e importanti, come quelli del settore della giustizia. Un chiaro esempio delle risposte mancate riguarda la questione del rinnovo contrattuale: con un'inflazione galoppante e una riduzione del potere d'acquisto, ci saremmo attesi che il Governo affrontasse con serietà le proposte per il rinnovo del contratto nazionale 2022-2024, già scaduto da oltre un anno. Invece, anche in questo caso, la strada intrapresa è quella di sottrarsi al confronto e ignorare la questione. L'ultimo rinnovo risale al 2021. Il Governo, inoltre, non vuole rimuovere i vincoli di spesa, sia per il salario accessorio sia per la valorizzazione delle professionalità. E tutto questo si ripercuote negativamente sulla qualità del lavoro della pubblica amministrazione. Anche i sindacati hanno chiesto misure sulla valorizzazione del personale, sulla necessità di aprire un confronto serio sull'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione. Ma puntualmente, anche in questo caso, vi state sottraendo. Questo provvedimento, però, sarà ricordato come il decreto contro la Corte dei conti. Con un emendamento, durante la discussione alla Camera, è stato modificato il testo, inserendo la norma che mina il lavoro della Corte dei conti sui progetti del PNRR, togliendo a un organo giudiziario indipendente, alla magistratura contabile, le funzioni di controllo sulla corretta attuazione del Piano. È ormai evidente che, all'interno del Governo e della maggioranza, le divisioni sul PNRR, dalla revisione dei progetti alla possibilità di non spendere tutte le risorse, siano insormontabili e abbiano portato a pericolosi ritardi. Invece di cambiare passo, il Governo ha individuato nella Corte dei conti il capro espiatorio. Mi dispiace, ma non è così che recuperiamo il grande ritardo sul PNRR. Noi abbiamo bisogno di assunzioni per gestire il PNRR e nel decreto non si accenna minimamente a superare, in termini legislativi, quei vincoli che ad oggi, siccome vengono ancora una volta confermati, di fatto impediranno agli enti locali alle Regioni, ai Comuni, alle Province, di assumere finalmente quelle professionalità indispensabili nella gestione del PNRR. È per questo che chiediamo, a tutto il Senato, alla Presidenza e al Governo, di rivedere alcune questioni. Noi riproporremo i nostri emendamenti, perché la pubblica amministrazione è bene comune, indispensabile a garantire i veri diritti di cittadinanza delle persone, ma anche la crescita di questo Paese. Così com'è indispensabile che la pubblica amministrazione sia in grado di gestire al meglio, nella qualità e nei tempi che devono dare garanzia, la gestione del PNRR.

Sappiamo bene che tale provvedimento mira a rafforzare la capacità amministrativa, a potenziare le strutture delle nostre pubbliche amministrazioni, anche e soprattutto in una logica di attuazione del PNRR. questo testo va oltre: ovvero mira a migliorare, in generale, tutto il funzionamento della macchina dello Stato, una macchina tanto complessa quanto indispensabile e affascinante al fine di renderla sempre più attrattiva, virtuosa e meno farraginosa. I molti anni di blocco del *turnover* e dei concorsi pubblici, dovuto all'eccessiva rigidità delle regole di bilancio, hanno comportato un forte depauperamento di competenze e professionalità nelle pubbliche amministrazioni, sia a livello nazionale che locale, impedendo peraltro a molti giovani l'accesso alla pubblica amministrazione. In questo senso, tante e numerose sono state le sollecitazioni da parte dell'ANCI, a livello nazionale, rispetto a tale Gli effetti di quanto detto si sono fatti sentire nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto nei settori tecnici degli enti locali, fondamentali per la progettazione delle opere pubbliche e per la redazione di bandi e gare. Solo negli ultimi anni, anche per i pensionamenti che maturavano, ci si è resi conto del grave problema che si era determinato, ovvero che non vi era un equilibrio tra ingressi e uscite. La novità piena di questa provvedimento è il cambio di visione, contrariamente a quanto si diceva prima, e di prospettiva nei confronti della pubblica amministrazione: non un peso da alleggerire, una sovrastruttura da rimuovere, ma uno dei pilastri portanti dello Stato. Il dato di fondo che va ripristinato è il principio costituzionale per cui alle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso. Passo ora a un altro tema, quello che in questi giorni è stato oggetto di polemiche da parte degli organi di stampa, di stampa, a proposito del controllo concomitante della Corte dei conti e dello scudo erariale. Diciamo subito che il Governo con questo emendamento aveva e ha l'obiettivo di rispondere a esigenze insopprimibili relative alla necessità di accelerare l'esecuzione dei progetti del PNRR e immagino che su questo tutte le forze politiche non possano che essere d'accordo. Con l'emendamento del Governo, infatti, la Camera ha escluso il controllo concomitante della Corte dei conti su piani, programmi e progetti previsti, al fine di velocizzare le procedure e non trovare ostacoli alla realizzazione delle opere che - come è noto - devono essere completate entro il 2026. prorogata fino al 30 giugno 2024 la disposizione del cosiddetto scudo erariale. Quanto alla norma sui controlli relativi al percorso di attuazione del PNRR - una norma fondamentale per la riuscita del Piano e che ha tanto agitato la stampa - l'articolo 1 non altera il sistema dei controlli sul PNRR che il nostro Paese deve garantire ai sensi del regolamento. Si tratta di un controllo allo stesso modo efficace ed in linea con il regolamento europeo che richiede agli Stati membri l'attivazione di controlli efficaci. In questo senso ci sono

A mio modestissimo e personale parere, con la Corte dei conti si deve sicuramente cooperare, tenendo ben in mente però che in ogni caso non è possibile ledere la riserva di amministrazione: collaborare sì, ma evitando l'eccesso di ingerenza nell'attività della pubblica amministrazione; controlli sì, ma non troppi e inefficaci. *(Applausi)*. Anche la cosiddetta norma sullo scudo erariale non rappresenta una novità: in pratica si tende a evitare che funzionari pubblici siano restii all'adozione celere di atti amministrativi, la cosiddetta paura della firma. La proroga al 2024 ci sembra quindi del tutto legittima. Il decreto-legge, inoltre, contiene alcune norme di grande interesse. C'è il tema delle infrazioni europee,

della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). La pubblica amministrazione ritorna centrale - come è giusto - nelle strategie di sviluppo della Nazione, per un Paese che deve rispondere e correre velocemente. In questo percorso la spinta può e deve venire anche da una macchina amministrativa rinnovata e solidale. Meritano quindi apprezzamento e sostegno le misure del Governo che hanno l'obiettivo di potenziare l'amministrazione pubblica con interventi tesi anche a incentivare il reclutamento dei giovani. Anche questo punto era nel programma ed è stato onorato dal Governo Meloni. formazione e l'aggiornamento del personale e, per non lasciare nessuno indietro, si promuove l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Tutto questo perché nessuno deve rimanere indietro e affinché tutti siano parte di una Nazione che sia orgogliosa di se stessa. incentivo all'assunzione di giovani laureati con contratto di apprendistato per trentasei mesi o, attraverso apposite convenzioni con le università, per studenti di età inferiore a ventiquattro anni. Anche questo era un impegno della campagna elettorale che è stato onorato da parte del Governo Meloni. Il decreto-legge

specialmente nei piccoli Comuni dove, grazie alla funzione e alle speciali e trasversali competenze e all'alta specializzazione di cui sono dotati, possono gestire anche i complessi processi e procedimenti per la realizzazione degli investimenti del PNRR. Con questo provvedimento si aggiungono sul piano normativo altre pietre nella ristrutturazione di una pubblica amministrazione di cui si riconosce la funzione fondamentale per la nuova Nazione e il suo sviluppo. Ma questo non basta se non è accompagnato da una svolta culturale sia interna che esterna alla pubblica amministrazione. Serve che la pubblica amministrazione riacquisti autorevolezza attraverso la certezza delle sue funzioni e dei suoi servizi. Serve innescare processi virtuosi di motivazione del personale, riconoscimento e valorizzazione del merito; creare condizioni e opportunità di crescita professionale all'interno della pubblica amministrazione. Serve che i pubblici dipendenti abbiano sempre più il senso del valore e dell'onore di essere al servizio della Nazione, come recita la nostra Costituzione. signor Presidente, con questo decreto-legge riusciamo a dare un sostanziale contributo al processo di ammodernamento del nostro Paese. E anche questo era un punto del nostro programma che stiamo onorando, che il Governo Meloni sta portando avanti e che oggi è riconosciuto dagli esperti e dai dati OCSE, che danno atto di ritmi di crescita molto superiori a quelli dell'economia occidentale e anche di Germania e Francia, nostri alleati europei ma anche nostri *competitor* commerciali. Questo Governo sta lavorando per portare le imprese a produrre sviluppo e occupazione il settore della pubblica amministrazione è un tassello fondamentale che dobbiamo valorizzare sempre di più. Con questo provvedimento, che mira al rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, facciamo quindi un grande passo in avanti; facciamo un ulteriore sforzo per presentare agli italiani il volto di uno Stato amico del quale ci si può fidare. *(Applausi)*.

Come si usa dire, è l'ennesima toppa che questo Governo ha voluto mettere a un problema che invece sarebbe stato importante risolvere davvero, con una programmazione seria di interventi, in particolare di fronte alle scadenze del PNRR e ai ritardi ormai conclamati nell'attuazione dei progetti. Avete approvato un decreto-legge che, nel titolo, promette di rafforzare la pubblica amministrazione, ma in questi giorni si parla di un altro decreto della pubblica amministrazione. Ci aspettavamo che metteste finalmente un freno alla precarietà imperante nel nostro Paese, che non è colpa di questo Governo, lo voglio sottolineare.

Di fronte al dato della precarietà, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, era necessario decidere di investire risorse necessarie a un piano straordinario di assunzioni per riempire le carenze di organico che esistono negli uffici della pubblica amministrazione stessa. Niente di tutto questo: avete - come dicevo prima - partorito un topolino, l'ennesimo decreto *omnibus*, che poi strada facendo avete riempito di altre cose. Prima di arrivare a dire di cosa l'avete riempito, vorrei sottolineare almeno due questioni che erano state solevate attraverso i nostri emendamenti e quelli di altri colleghi dell'opposizione, ma che non hanno trovato alcun accoglimento, facendoci comprendere come vi sia una distanza ormai evidente tra chi governa il Paese e gran parte delle questioni concrete e reali che riguardano la vita delle persone. Mi riferisco, ad esempio, alle attese e alle legittime aspettative che da anni nutrono i lavoratori e le lavoratrici impegnati a rendere efficiente il sistema giudiziario del nostro Paese. In particolare mi riferisco agli addetti all'ufficio per il processo,

per far fruttare l'investimento che la pubblica amministrazione ha fatto nel formarli. E invece no: li formiamo per mesi, li mettiamo a lavorare e poi decidiamo di mandarli a casa. È inutile che stia a dirvi in quali condizioni sono i nostri tribunali e a rammentarvi le condanne dell'Italia per l'eccessiva lunghezza dei processi. Eppure, non ci curiamo degli addetti ai processi e allo stesso tempo consentiamo di declassare a semplici funzionari coloro che rivestono da anni posizioni giuridiche di direttore, in virtù delle quali sono stati conferiti deleghe e incarichi di elevata autonomia e responsabilità.

a risolvere almeno qualche questione. C'è poi un'altra questione che voglio sottolineare. Pensiamo ai lavoratori e ai docenti dell'AFAM: in migliaia hanno chiesto, a differenza di ciò che è avvenuto, un intervento puntuale e mirato che potesse risolvere il loro problema

una doppia procedura per l'immissione in ruolo dei docenti che, dopo tre anni di servizio come docenti AFAM, avrebbero la possibilità di partecipare al concorso straordinario per

La Corte dei conti ha evidenziato dei ritardi nella realizzazione del PNRR, facendo presente che certi ritardi a volte sono colpevoli e quindi sanzionabili. Voi cosa avete fatto? Avete presentato di notte un emendamento proprio sulla Corte dei conti per limitare il controllo che la legge gli conferisce sul PNRR. Questo è quanto avete fatto. Quindi a un certo punto è arrivato alla Camera l'emendamento che eliminava tale misura. Credo invece che abbiamo la necessità di partire da quanto invece ha detto il presidente della Corte dei conti in una audizione definita informale, ma ottenuta solamente grazie alla richiesta delle opposizioni. In quella occasione il presidente Carlino ci ha detto che il controllo concomitante non è la causa dei ritardi del PNRR, ma al contrario accelera e migliora la qualità del procedimento amministrativo.

sia controllato dalla Corte dei conti. Si vuole accentrare il potere, e questo ve l'ho già detto. C'è una concezione in questa maggioranza che mira a portare tutto al centro, in particolare alla Presidenza del Consiglio, e dà molto

dobbiamo stare molto attenti, perché in questo Paese abbiamo avuto esperienze molto negative: se si allargano le maglie del controllo, c'è il rischio di infiltrazione mafiosa e,

che hanno studiato e che hanno lavorato da precari negli uffici della pubblica amministrazione. La sfida del PNRR è epocale e richiede una pubblica amministrazione efficiente, in grado di affrontare tali questioni. Per questo motivo e soprattutto per quanto detto all'inizio del mio intervento, e cioè per l'incapacità totale di questo provvedimento di affrontare concretamente i problemi del Paese e di dare una risposta concreta a tanti lavoratori e lavoratrici, il nostro giudizio è fortemente negativo. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, con questo provvedimento forse, così come preannunciato, saremo davanti alla diciottesima questione di fiducia posta dall'insediamento di questo Governo. In otto mesi, diciotto fiducie sono state poste per sancire non solo la scomparsa del dibattito parlamentare, così come richiamato dal presidente della Camera Fontana, ma anche e soprattutto la farsa della coesione della maggioranza che sostiene questo Governo. Onorevoli membri del Governo, la fiducia, se la porrete, non la imponente a noi dell'opposizione: la fiducia la state imponendo ai vostri parlamentari. Tra l'altro, state dimostrando e state mostrando agli italiani ciò che veramente siete:

ha occupato tutti i posti del potere; una destra che, dove non può arrivare piazzando i propri uomini di fiducia - così come è avvenuto e come avviene nelle autorità di controllo indipendenti tenta di azzittirli a colpi di sconcertanti interventi normativi. La cosa però più amara da constatare è che, nonostante questa prova di forza, con questo provvedimento non ci sarà alcun rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Il piano di assunzioni proposto è inadeguato alle richieste di rinnovamento delle nostre pubbliche amministrazioni e insufficiente a colmare il *gap* dovuto alla dinamica dei pensionamenti. Il provvedimento in esame si concentra esclusivamente sul riassetto dei vertici, tralasciando, forse appositamente, il vero cuore e il vero problema della pubblica amministrazione: il reclutamento di nuove e maggiori competenze professionali e tecniche. Non c'è alcuna azione per potenziare la pubblica amministrazione; alcuna proposta per potenziare l'efficienza dei servizi ai cittadini. È stata, questa, una scelta voluta dal Governo. Diciamocelo chiaramente, colleghi: se la pubblica amministrazione funzionasse davvero, il Governo non avrebbe alcuna scusa per scaricare le responsabilità della spesa, anzi della non spesa dei fondi europei sugli enti regionali e sugli enti locali. Può quindi sorprenderci la proroga fino al 30 giugno 2024 dello scudo erariale per i dirigenti di Stato? Lo sappiamo tutti: le condizioni sono mutate e non c'era alcun motivo per prorogarlo, a meno che l'obiettivo del Governo non era proprio impedire di perseguire i responsabili del danno erariale o impedire di recuperare le somme distratte. Ma questo non vi è bastato. Nello stesso emendamento governativo vi è stato anche il tentativo di imbavagliare la Corte dei conti sull'attuazione del PNRR tentativo in parte fallito, così come ci rassicura il Presidente della Corte dei conti, che ha dichiarato, in occasione del convegno dell'università Cattolica di Milano, di Milano, citato dall'onorevole Melchiorre, che il controllo sulla gestione e dunque anche il controllo in corso d'opera, cioè il controllo concomitante, è principio incomprimibile garantito dalla nostra Costituzione all'articolo 100. Pertanto, nonostante l'azione del Governo, il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti potrà essere effettuato e noi non possiamo che essere confortati da questa affermazione. Ma resta il fatto che ci avete provato e già questo basta a preoccuparci e dovrebbe preoccupare tutti tutti i presenti in quest'Aula, perché non c'è alcun atto, alcun documento, alcuna analisi che attesti che il controllo concomitante rallenti l'attuazione dei progetti all'interno del PNRR. Allora, colleghi, mi chiedo e domando anche a voi: qual è stata la *ratio* del Governo? Governo? L'unica risposta che ho trovato possibile è proprio il tentativo di limitare il controllo della Corte dei conti. E questo è molto pericoloso, colleghi, perché certifica la delegittimazione da parte del Governo del ruolo fondamentale delle autorità di controllo indipendenti, dell'equilibrio tra controllori e controllati, dell'equilibrio tra sistemi di gestione e sistemi di controllo, la cui assenza svuota di significato la parola democrazia. Parliamoci chiaramente: cosa ha fatto di così grave la Corte dei conti? Ha solo certificato ciò che è sotto gli occhi di tutti, ossia il gravissimo ritardo nell'attuazione del PNRR. Il Governo Meloni ha speso appena un miliardo sui 33 miliardi previsti dal Piano per il 2023. Forse, colleghi, non ve ne siete accorti, ma siamo già a giugno 2023. La settimana scorsa sono arrivati gli ispettori della Commissione europea, per una visita di *routine* - è vero - che fanno dappertutto; l'hanno fatta in tutti i Paesi che hanno beneficiato e beneficiano del PNRR.

di ciò che sta accadendo nella rimodulazione del PNRR. Come all'oscuro è anche il Parlamento: noi non sappiamo quali sono i progetti che verranno definanziati perché non realizzabili. Questo non è corretto, perché perché non è possibile che il Parlamento, le parti sociali e tutta la la società italiana non vengano coinvolti in questa grande sfida. sfida. Consideriamo poi un altro aspetto. La visita degli ispettori - come abbiamo appreso dagli organi di stampa - ha certificato le tensioni interne a queste Esecutivo: tra il Ministero guidato dal ministro Fitto e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha rivisto previsioni e cancellato interi passaggi sulla stima finanziaria del *recovery*; e quelle interne al Ministero delle infrastrutture, che vuole procedere alla riallocazione automatica dei fondi inutilizzabili. Il tutto mentre ancora stiamo aspettando l'erogazione della terza rata. *(Applausi)*. Non sappiamo neanche quando sarà fatta la richiesta della quarta rata.

che a giorni arriverà l'erogazione della terza rata. E meno male, io dico. Forse, colleghi della maggioranza, non vi siete resi conto e vi siete scordati che la richiesta dell'erogazione della terza rata è avvenuta a dicembre 2022; siamo a giugno 2023, termine della scadenza

le richieste di erogazione delle rate secondo il calendario predisposto dal Piano - come hanno fatto tanti altri Paesi europei - noi possiamo anche chiederle dopo. Forse però il ministro Fitto non ricorda che l'Italia è in una condizione economico-finanziaria diversa dagli altri Stati d'Europa: se noi abbiamo avuto il PNRR più corposo, è proprio perché dovevamo superare tanti divari. Lo dice l'Istat, non lo diciamo noi: senza il PNRR l'Italia già quest'anno sarebbe in stagnazione. Signor Presidente - e mi accingo a concludere - noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo cercato con i nostri emendamenti e i nostri ordini al giorno di difendere giustizia e buonsenso. Ribadiamo la completa disponibilità a collaborare per non perdere neanche un euro del PNRR. Ancora una volta chiediamo al Governo di investire tutti i fondi che non è in grado di spendere su Transizione 4.0 e superbonus; tra l'altro - com'è stato affermato dall'Esecutivo nella relazione - il tasso di spesa è superiore al 60 per cento. Ripensate a quello che fate e agite in nome e per conto di tutti gli italiani e, soprattutto, ricordate che gli italiani hanno pagato un costo altissimo per avere un Paese democratico e pertanto abbiatene rispetto.

devo ammettere che oggi ho qualche difficoltà a intervenire in quest'Aula senza sentire l'esigenza di manifestare un profondo malessere. Avverto forti su di me le conseguenze che derivano - da un lato - da un ricorso sempre più comune alla decretazione d'urgenza e - dall'altro lato - dalla conseguente compressione dei lavori parlamentari. Nonostante sia la mia prima esperienza parlamentare, so benissimo che queste dinamiche hanno accomunato le forze politiche che oggi siedono ai banchi dell'opposizione e che ieri erano tra quelli della maggioranza. Osservo con grande preoccupazione che, se ogni Governo che arriva fa peggio di quello che lo ha preceduto e non prova a fare lo sforzo di ristabilire una certa normalità nel procedimento legislativo, si corre il rischio di distorcere il nostro sistema istituzionale. Questa è una preoccupazione della quale noi tutti, a prescindere dal fatto di svolgere il ruolo di maggioranza o opposizione, dovremmo farci carico. carico. Tutti noi dobbiamo avere cura della nostra democrazia: la democrazia non è una cosa che si conquista una volta per tutte; va manutenuta, protetta e rafforzata ogni giorno, con l'impegno di tutti. Fino ad oggi questo Governo ha approvato una media di più di quattro decreti al mese. Parliamo di un Governo che si è appena insediato e che supera immediatamente la media dei Governi precedenti. Con questi numeri il presidente Meloni, dall'opposizione, avrebbe pronunciato esattamente le mie parole, magari con un po' più di enfatizzazione, ma ognuno del resto ha il suo stile. Se poi penso che questo decreto è stato il primo approvato dai colleghi deputati, dopo l'incontro tra i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente della Repubblica, in cui lo stesso Presidente ha sollevato la criticità legata al fatto che l'attività parlamentare avviene esclusivamente attraverso decreti-legge e che oltretutto su quasi la totalità di questi decreti viene posta la questione di fiducia, capite bene che la preoccupazione non può che aumentare. Mi auguro - e su questo faccio appello anche alla Presidenza - che queste Aule possano tornare finalmente a lavorare, così come avevano previsto i Padri costituenti, con dignità, competenza e rispetto dei ruoli. Venendo al merito del decreto, il titolo poteva davvero lasciar sperare che si affrontasse una questione centrale come lo stato di salute, l'organizzazione e il potenziamento della macchina amministrativa dello Stato. È stato invece partorito un topolino, al punto che a questo decreto il Governo ne ha fatto subito seguire un altro: un decreto pubblica amministrazione-*bis*, che altro non fa che darci la cifra di come il Governo abbia agito, senza una visione complessiva e senza l'intento di attuare una vera riforma in grado di rilanciare la pubblica amministrazione. Ha piuttosto approvato provvedimenti spezzatino, che sembrano quasi

Le amministrazioni italiane hanno perso oltre 213.000 impiegati a tempo pieno dal 2008 al 2021. Stiamo parlando di numeri importanti che mettono a rischio il funzionamento delle stesse nostre amministrazioni. Le difficoltà sembrano essere già evidenti in relazione all'applicazione e alla messa in atto del PNRR. Mancano figure sulle quali i nostri Comuni e gli enti locali, prossimi al cittadino, possano contare. Ecco perché questo provvedimento poteva e doveva essere una grande opportunità per il nostro Paese. Ecco perché penso che insieme avremmo dovuto fare uno sforzo per potenziare la macchina amministrativa degli enti pubblici, a cominciare dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato centrale, investendo di più sul personale, su forze fresche, sui lavoratori più qualificati, maggiori competenze e conoscenze. Ritorno sul PNRR, e non solo per ribadire un concetto che trovo fondamentale: il PNRR è una grandissima opportunità per il nostro Paese. Questa discussione sulle modifiche o sull'opportunità di usare o meno determinate risorse del Piano è fuori da qualsiasi logica. Noi dobbiamo preoccuparci di una sola cosa: spendere quei soldi, spenderli bene e spenderli in tempo. Tutto il resto rientra in una discussione che può solo danneggiare l'Italia. Ed è per questo che il tentativo che sta portando avanti il Governo con questo decreto è gravissimo. Togliere alla Corte dei conti la possibilità di un controllo sui fondi PNRR è un fatto che si commenta da da sé e che rischia di creare un precedente gravissimo. E anche qui torno al merito. Il Governo, alla Camera dei deputati, aveva inserito, tramite emendamenti, due questioni che nulla avevano a che vedere con l'oggetto originario del decreto-legge: uno riguardante il Ministero della difesa, poi fortunatamente ritirato, e uno che rivede le prerogative di un organo importantissimo come la Corte dei conti. Onorevoli colleghi, non so se vi rendete conto di quanto possa essere grave non solo il merito della questione, ma anche il metodo che avete usato. Ma di cosa avete paura? Perché intervenire sul cosiddetto controllo concomitante? Voglio solo ricordare ricordare che il controllo concomitante - esattamente come ha detto il presidente della Corte dei conti, Carlino - «ha la finalità specifica di accelerare gli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, ha una funzione propulsiva» non di ostacolo «in esito alla quale l'amministrazione può porre in essere percorsi autocorrettivi». Voi invece interpretate questo controllo come un ostacolo e dunque prorogate lo scudo ed eliminate il controllo. Il risultato è che stiamo di fatto smontando un sistema di controlli costruito a garanzia dei cittadini e anche Fa abbastanza sorridere, inoltre, che nella scorsa legislatura fossero state proprio le forze di opposizione a chiedere, con una proposta di natura parlamentare, che venissero aumentati i controlli della Corte dei conti sul PNRR. Vi è bastato andare al Governo per cambiare idea, in modo diametralmente opposto. *(Applausi)*. Capiamoci: non ci stupisce che possiate aver cambiato idea; ce ne siamo fatti abbastanza una ragione. È che cambiarla così velocemente, con convinzioni opposte, lascia abbastanza spiazzati, per usare un eufemismo. Infine, signor Presidente, vorrei far presente il seguente dato e i seguenti numeri: 300.000 persone andranno in pensione nel 2026, 700.000 nel 2030, e ciò solo nella pubblica amministrazione e nella sanità, senza considerare la scuola e l'università. Parliamo di comparti fondamentali per il nostro Paese: servizi di prossimità, di cura, di educazione dei nostri cittadini.

così complesso, di natura sistemica, il provvedimento che stiamo discutendo rischia di coprire di ridicolo finanche il nostro impegno politico e la credibilità delle cariche che ricopriamo. allora un serio appello al Governo e alla maggioranza: lavoriamo affinché possano saltare una volta per tutte i tetti alle assunzioni delle pubbliche amministrazioni. Diamo la possibilità di stabilizzare, ad esempio, i circa 63.000 medici precari. Rivediamo insieme gli stipendi di tutto il personale sanitario. Partiamo da qui, ma con un processo di riforma serio e completo. In questo provvedimento non c'è niente di tutto ciò: manca una visione di sistema; manca una riforma organica della pubblica amministrazione; mancano le risorse per assumere e rafforzare la Peccato che invece ci sia l'ennesimo schiaffo alla trasparenza e ai controlli. Questo Paese merita altro, meritiamo di meglio dell'ennesimo provvedimento senza forza, visione e strategia.

prevede disposizioni urgenti per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, al fine di dare finalmente risposte giuste ed efficaci alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di essere all'altezza, in termini di operatività ed efficienza, nell'attuare un piano straordinario come il PNRR, che prevede complesse procedure di gestione. Per questo, mai come ora, era necessario dotare le amministrazioni di risorse umane e competenze di eccellenza, per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, così come era impensabile non attuare il più grande investimento di riforme e di risorse per l'ammodernamento del nostro Paese, caratterizzato da organici che hanno risentito del blocco del *turnover* per svariati anni. Infatti, a partire dal 2018, le assunzioni nella pubblica amministrazione sono state bloccate attraverso una serie di provvedimenti che hanno previsto anche limitazioni alla sostituzione del personale in uscita, rendendo ancora più drammatica la situazione nei piccoli Comuni, dove la copertura di un solo dipendente rappresenta un problema insormontabile, del progressivo invecchiamento del personale, scarsamente aggiornato, rendendo così la pubblica amministrazione fragile e, in molti casi, incapace di offrire servizi adeguati a imprese e cittadini. Da qui, quindi, l'esigenza di potenziare e stabilizzare gli organici, per evitare il rischio di una paralisi dell'ordinaria amministrazione, in vista anche dei grandi impegni che gravano sui piccoli Comuni e sulle realtà territoriali, enti attuatori del PNRR, ma soprattutto di garantire il futuro della nostra Nazione, considerato che una pubblica amministrazione moderna ed efficiente è sinonimo di sviluppo di un Paese. In quest'ottica va la previsione di alcuni interventi, come la stabilizzazione dei dipendenti che hanno lavorato per almeno tre anni presso uffici di Regione, Provincia e Comuni, la stabilizzazione del personale impiegato negli uffici speciali per la ricostruzione del post-sisma e la possibilità, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di assumere in via definitiva i segretari comunali, assicurando loro una figura professionale indispensabile all'attività amministrativa, soprattutto in attuazione del PNRR. Altro intervento importante previsto nel provvedimento è quello di innalzare al 12 per cento, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione, incarichi dirigenziali in amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per l'attuazione del PNRR. Si è previsto l'ampliamento degli organici del comparto difesa e sicurezza, comprendendo naturalmente le Forze armate, Carabinieri, Polizia, Capitaneria di porto e Vigili del fuoco, con 2.100 assunzioni. Una svolta storica è rappresentata dall'inserimento della carriera dei medici nel Corpo di polizia penitenziaria, visto che questa era l'unica, tra le forze di polizia, a non essere dotata di questo ruolo tecnico. Queste sono risposte vere e concrete, da parte di un Governo che, attraverso interventi fondamentali, vuole supportare tutti gli uomini e le donne che quotidianamente, con il loro servizio, garantiscono la sicurezza dei cittadini, il territorio, la prevenzione, il contrasto della criminalità e di attività terroristiche. Tale Governo ha ugualmente l'obiettivo di dare valore alle professionalità e alle eccellenze: non come i passati Governi, che hanno tagliato unilateralmente organici, provveditorati regionali e scuole di formazione! Rispetto alla scuola, è stata prevista per i dirigenti scolastici la mobilità, per l'anno scolastico 2023-24, sul 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna Regione, sbloccando così la grave situazione di disagio cui sono soggetti numerosi dirigenti collocati fuori Regione. È prevista inoltre la proroga di un anno del vincolo triennale di mobilità per i docenti neoassunti in ruolo, che permette a tanti docenti di ricongiungersi finalmente alle loro famiglie. Con un emendamento di Fratelli d'Italia sono poi stati reintegrati nel posto di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023, i dirigenti scolastici licenziati assunti con riserva. E per garantire l'inclusione nelle comunità scolastiche si è intervenuto in modo concreto sul sostegno, prevedendo lo scorrimento delle GPS di prima fascia, sostegno ed elenco aggiuntivo. E se dovessero residuare ancora posti, si procederà ad una mini*-call* veloce. Infine, alle tante polemiche assolutamente strumentali su un emendamento governativo che prevedeva la proroga delle limitazioni della responsabilità contabile, rilevo

oggi, in un momento in cui ci sono tempi ristrettissimi e bisogna portare a compimento un piano poderoso e complicato come il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una norma del genere appare più che mai necessaria. Per non parlare poi del controllo concomitante: ancora attacchi fuorvianti da chi ha solo l'obiettivo di screditare un Governo che sta lavorando per attuare quanto previsto nel PNRR. Non c'è nessun tentativo di privare la Corte dei conti del suo potere; non è così, come ha detto lo stesso Presidente della Corte dei conti, affermando che disciplinare le modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti è nella piena legittimazione del Governo e del Parlamento. Diciamo quindi forte e chiaro che il controllo contabile sul PNRR non è stato affatto soppresso; il controllo c'è, ma si svolge nelle forme del controllo successivo di gestione a criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea. Rispetto poi alle catastrofi preannunciate e alle innumerevoli critiche strumentali di chi vuole nascondere il proprio fallimento di questi anni, rispondiamo che negli ultimi mesi l'economia italiana è cresciuta e continua a crescere più del previsto nel primo trimestre del 2023 il PIL italiano è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,9 per cento nei confronti del primo trimestre del 2022, un incremento superiore a quello di Francia e Germania. I dati diffusi dall'Istat dimostrano chiaramente che gli occupati sono cresciuti di oltre mezzo milione rispetto al primo trimestre del 2022. Questi sono dati inconfutabili, che confermano ancora una volta che questo è il Governo del fare, che lavora per il benessere dell'Italia, per ridare slancio all'economia nazionale, per costruire una Nazione più dinamica, competitiva e al passo con le sfide del nostro Paese.

signor Presidente. Con il reddito di cittadinanza si permettono di aizzare odio contro un Governo che in pochi mesi è stato capace di dare risposte serie e concrete ai cittadini Mi riferisco in modo particolare, signor Presidente, al signor Grillo che, per avere un momento di gloria, visto che era del tutto scomparso dalla scena politica, ha usato parole pesantissime, che evocano un passato oscuro per la nostra Nazione, promuovendo lavoro gratuito, illegale e rischioso, un vero insulto alle continue battaglie per ottenere maggiore sicurezza sul lavoro; un vero insulto alle tante famiglie che ancora oggi piangono e hanno la morte nel cuore per i loro cari morti sul lavoro. lavoro. Tutto ciò è veramente inaccettabile e ancora più inaccettabile è il tentativo di minimizzare l'accaduto. Oggi qualcuno dovrebbe chiedere scusa agli italiani che hanno riconosciuto il lavoro fin qui svolto da questo Governo e che non si lasciano abbindolare da questi imbonitori di piazza, gente che non sa più che farsene degli insulti e delle cattiverie e delle cattiverie gratuite, che disdegna e disprezza. Rassegnatevi, non sarà il vostro odio a distruggere il consenso che abbiamo costruito dando risposte serie e concrete agli italiani.

della direzione nazionale del Partito Democratico, un evento importante in modo particolare - mi rendo conto - per i senatori e le senatrici del Partito Democratico.

Nel dibattito poi si esprimono opinioni che non sempre sono apprezzate dagli uni o dagli altri; è per questo che c'è una pluralità di voci e la Presidenza interviene quando si superino dei limiti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei pensato di chiedere la parola in quest'Aula per portare il nostro saluto istituzionale a un uomo come Nuccio Ordine, uomo di lettere, uomo di cultura *tout court*, professore all'Università della Calabria ma *visiting professor* nei più importanti atenei del mondo, da Yale alla Sorbona, accademico di fama mondiale, membro del Comitato scientifico della Treccani, insignito di numerose lauree *ad honorem* e di importantissimi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui - ultimo in ordine di tempo

Mirabilissimi i suoi studi sul Rinascimento, su Steiner, su Giordano Bruno, di cui era considerato uno dei massimi esperti. Il *fil rouge* che collega tutta l'opera di Nuccio Ordine si esplica nel suo celeberrimo manifesto dal titolo «L'utilità dell'inutile», assurto a *bestseller* mondiale, tradotto in oltre trenta lingue, in cui in maniera molto concisa sottende l'importanza della memoria. Mnemosine, la memoria, è divinizzata e venerata; sono le muse, sue figlie, a presiedere le esperienze intellettuali e artistiche, ma qual è l'esperienza decisiva di conoscenza? Aristosseno di Taranto e Platone propendono per la memoria che, assieme alla filosofia, consentirà all'uomo di essere degno di salire sulle stelle. Ernst Bloch definisce lo spazio della morte come spazio dell'invisibile in cui inizia e verso cui seguita a tendere un universo finalmente senza più esteriorità in quanto prevale in lui la verità. Nel lavoro di Nuccio Ordine nulla è finzione, ma pure si incastra entro una storia in cui i maestri di pensiero sono i protagonisti ed è mirabile davvero quanto l'autore sappia quasi rimanere discretamente da parte affidandosi a loro con una formidabile capacità di coglierne l'essenza. Un intellettuale legato alla terra della Calabria, quella Magna Grecia che ricollega Nuccio Ordine all'archetipo stesso della nostra cultura, la letteratura europea

una lucidissima analisi del *hic et nunc* che egli proponeva attraverso la lettura dei grandi classici. Emergeva nel suo pensiero quanto anche la sapienza e non il sapere fine a sé stesso, ma pure la bellezza o l'estetica necessitino per essere comprese di una partecipazione appassionata,

Per il professor Ordine l'importanza dello studio era fonte di conoscenza; da qui la necessità che lo studio sia accessibile a tutti. La sua vita era segnata dalla passione e dall'impegno. Ciò ci porta a riflettere su quale forza rappresenti la conoscenza, che sempre i regimi totalitari hanno cercato di limitare. Si dominano gli ignoranti dunque, ma se sono gli ignoranti a voler dominare, l'umanità stessa rischia di estinguersi e di essere repressa. Nell'opera di Nuccio Ordine però anche sempre il presente, la *dignitas* *hominis* che una società con una scala gerarchica di valori completamente stravolta ha perduto per cedere il passo a volte alla prostituzione della sapienza. Nuccio Ordine è stato letterato, ma anche filosofo. Le riflessioni su Giordano Bruno toccano il tema della libertà e definiscono il *nonsense*. Ricordo però anche il suo saggio su Enrico III, il sovrano francese che si adoperò far cessare le guerre religiose. Nuccio Ordine ha voluto dare senso alla cultura umanistica anche con la scelta di essere tra i soci fondatori, con Umberto Eco e Elisabetta Sgarbi, della casa editrice La Nave di Teseo. Mi piace, in conclusione, citare una frase che che Nuccio Ordine ha proferito in occasione del suo discorso per il conferimento dell'onorificenza francese di cavaliere dell'Ordine delle Palme accademiche: solo chi si libera dei propri egoismi personali può intraprendere il difficile e gioioso cammino della conoscenza. Alla famiglia, agli amici e ai suoi studenti il nostro pensiero commosso. Buon viaggio professor Ordine. Ciao Nuccio. Presidente, mi rivolgo a lei per parlare al Governo, ai colleghi del centrodestra e soprattutto ai cittadini fuori che stanno guardando quello che succede sul tema dell'alluvione in Emilia-Romagna.

Io non so cosa stia succedendo. Spero - mi auguro - che non sia una brutta parentesi politica sul nostro territorio, sulle spalle delle persone.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

La seduta è tolta